Colleghi, è presente in tribuna una delegazione della Commissione integrazione europea del Parlamento croato, guidata dal suo presidente, in visita ufficiale al Senato su invito della presidente della Commissione politiche dell'Unione europea, senatrice Boldi.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 13.700 (già 2.218), 46.900, 47.1000/2, 64.700 e 66.0.700, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 13.700. In relazione alle proposte 64.700 e 66.0.700 ribadisce parere non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la parola "possono" sia sostituita dalla parola "devono". In relazione infine all'emendamento 46.900, ribadisce la condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, già espressa sul testo nel parere del 27 aprile 2010, volta ad inserire in fine il seguente periodo: "I costi per l'espletamento delle procedure concorsuali devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti". Ove tale condizione non fosse accolta, il parere si intende contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'articolo 47 del testo. Il parere di nulla osta sul subemendamento 47.1000/2 è dato quindi nel presupposto dell'accoglimento della condizione di cui sopra».

la rappresentante del Governo mi ha gentilmente fornito questa mattina i dati sulla consistenza del partito degli avvocati in Senato: 44 senatori, più del 13 di quest'Assemblea. Siamo sostanzialmente il terzo partito, con una netta sovrarappresentazione

i giovani, i collaboratori, in particolare coloro che, senza essere titolari di studio, lavorano a tempo indeterminato e continuativo per un unico studio.

circa 50.000; dato confermato, anzi aumentato, dalla Cassa di previdenza degli avvocati. Sono avvocati sostanzialmente a stipendio. In questa legge,

del rapporto di lavoro autonomo, si toglie a questi 50.000 avvocati dipendenti l'autonomia sostanziale. Questi collaboratori possono essere licenziati da un giorno all'altro, senza un minimo di preavviso e anche per il motivo più futile. L'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato per loro non esistono. Si finge che siano autonomi, in realtà dipendono a tutti gli effetti dal loro *dominus*, dal titolare dello studio. Se si ammalano, gli studi seri li sostengono, mentre gli studi meno seri li lasciano senza una lira di sostegno del reddito. delle malattie consistenti, di quelle che possono comportare l'interruzione del lavoro per mesi e quindi incidere notevolmente sulla loro condizione.

fatto che i Consigli dell'ordine, applicando una norma come questa, non hanno mai cancellato dall'albo i 50.000 dipendenti a tempo indeterminato in condizione di monocommittenza e di sostanziale dipendenza.

proporre in Commissione, senza che ci sia stata data una parola di risposta, non è stato certo di trasferire su questo rapporto l'intero diritto del lavoro subordinato: sappiamo che questo non avrebbe senso. Occorre però riconoscere

riconoscendo la particolarità di questo rapporto di dipendenza e provvedendo di conseguenza con una normativa speciale, disegnata in funzione di questo rapporto particolare. È esattamente la stessa cosa che è stata fatta nel 1981 per i calciatori e gli atleti professionisti, cui si è riconosciuto, a determinate condizioni, il carattere di lavoratori dipendenti, dettando però una disciplina adatta Non lo volete fare? dall'albo di 50.000 nostri collaboratori, che oggi lavorano in condizione di sostanziale subordinazione, anche se negata dalla legge.

dall'entrata in vigore della presente legge, ad opera del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dei criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali tra committente e collaboratore. Questi erano stati i rilievi

in via generale ha le sue caratteristiche; se si instaura tra due avvocati, uno anziano e uno giovane, invece, cambia totalmente. Se si svolge un'attività di lavoro subordinato attraverso la prestazione di opera professionale presso uno studio legale, esso non viene qualificato per legge come rapporto di lavoro subordinato e non è sottoposto alle regole e alla tutela per il contraente più debole, che nel caso di specie è il giovane avvocato

di incostituzionalità che una norma di questo tipo può avere, non capisco la ragione per la quale non si acceda alla tesi sostenuta nell'emendamento successivo,

che si svolge secondo le regole dell'attività libero professionale e che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato perché ciò crea una serie di problemi, un altro conto sono tutte quelle altre prestazioni di attività professionale che vengono rese nella sostanza e nella forma di un rapporto di lavoro subordinato all'interno dei grandi studi legali e che, in base a tale disposizione, non trovano alcuna tutela.

Presidente, il tema è meritevole e mi fa piacere che adesso tutti lo riconoscano. Abbiamo fatto una serie di formulazioni di questo

siamo giunti alla determinazione di non poterlo approvare perché si sarebbe creata una situazione particolare e complessa, una sorta di riserva, pur comprendendo le ragioni che sono

*(PD)*. Vorrei sottolineare che questa rinnovata contrarietà del relatore e del Governo all'emendamento 15.205 contrasta con le conclusioni del dibattito che si svolse su questo emendamento nella seduta dell'altra settimana, allorquando, di fronte all'evidenza di taluni argomenti che venivano espressi, era stata dichiarata una disponibilità, magari anche riformulando il testo, ad accogliere una norma di questo tipo. Io credo che la posizione della maggioranza sia sbagliata e grave, e vorrei che i colleghi si rendessero conto di quello che stiamo decidendo. In sostanza, per i reati minori

per lo più di persone che non possono permettersi la nomina di un difensore di fiducia o che vivono una condizione di disagio, di emarginazione o altro, viene svolta dagli avvocati che hanno meno da fare, diciamo così, da quelli che vivono una condizione - purtroppo - di marginalità professionale. E se qualche avvocato affermato si candida a svolgere queste attività per lo più delega il giovane di studio, delega il praticante, delega chi può. Con il testo dell'articolo 15, noi, stabiliamo

accumulato un certo numero di anni. Il senatore Valentino, nella seduta in cui abbiamo discusso di questo testo, ebbe a dire che anche davanti al giudice di pace dobbiamo garantire il massimo della professionalità, perché anche la difesa d'ufficio è un'attività tale per cui va garantito il massimo di professionalità, in tal modo formulando un un auspicio che è contrarissimo a quello che avviene tutti i giorni negli uffici giudiziari italiani: non c'è un avvocato affermato che vada a fare la difesa d'ufficio. Nessuno: sfido chiunque a dimostrare il contrario.

questo riflettere seriamente e fare in modo che la difesa d'ufficio davanti al giudice di pace, davanti ai tribunali, per i reati che erano di competenza della pretura, venga garantita prioritariamente ai giovani? Neanche questo. Non capisco quale sia l'impedimento procedimentale, quali problemi si creerebbero, quale stravolgimento del testo si determinerebbe. Noi potremmo stabilire con una norma semplice che alcune decine di migliaia di procedimenti se li fanno i giovani, quelli ai quali nessuno pensa; davvero non capisco quale sia la ragione di questa contrarietà. Per questo non mi rassegno alla cecità della maggioranza e del Governo e chiedo ai colleghi di riflettere e di votare a favore abbiamo discusso a lungo in Commissione e si era evidenziata la necessità di un aggiustamento tecnico.

che siano iscritti all'albo da non più di sei anni: quindi, da sei anni e un giorno non si può assumere la difesa. Il comma che precede stabilisce che per essere iscritti nell'albo bisogna avere però un altro titolo, quello di cinque anni precedenti l'iscrizione senza avere riportato sanzioni disciplinari. Il combinato di questa disciplina comporta che esclusivamente gli iscritti dal quinto al sesto anno possono assumere la difesa: i primi cinque anni una condizione di iscrizione, perché per cinque anni non bisogna avere riportato sanzioni disciplinari; possono essere nominati quelli che hanno una iscrizione inferiore a sei anni; sei anni meno cinque fa un anno. si determinerebbe una specie di riserva indiana per cui solo gli avvocati iscritti dal quinto al sesto anno potrebbero assumere le difese così come previste nell'emendamento.

creerebbe veramente grande confusione. Altro che migliaia di giovani avviati alle difese d'ufficio: sarebbe uno spicchio

Presidente, signore e signori del Senato, vorrei ricordare al senatore Legnini, e anche al senatore Li Gotti, la sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2010. Si è parlato qui diffusamente dell'apertura che si doveva dare ai giovani più deboli, evidentemente questo argomento non è stato ritenuto sufficiente dalla Corte costituzionale, che ha stabilito che i praticanti avvocati abilitati - dopo un anno sappiamo che possono essere abilitati non possono essere difensori d'ufficio; possono invece essere difensori di fiducia. L'argomento, un po' brutale nella sua sintesi (con il massimo rispetto per la Corte costituzionale), sul punto "né può costituire argomento contrario la possibilità, per il praticante avvocato, di essere nominato difensore di fiducia: un conto è che tali limiti di competenza professionale e di capacità processuale siano liberamente accettati dall'imputato,

grande forza alla difesa d'ufficio ma si è contemporaneamente detto che questa deve essere attuata soltanto da professionisti di pieno diritto, cioè non dai praticanti avvocati che hanno il patrocinio. La logica dell'articolo 15 è in questa linea: a regime, la difesa d'ufficio dovrà essere attuata semplicemente e solo dagli avvocati specialisti in diritto penale; allora creare una norma di carattere transitorio (e si potrebbe capire che nel periodo transitorio si possa avere un disciplina diversa e, essendo una norma transitoria, sappiamo che la Corte costituzionale

diversi sulle quali intendo prendere posizione. Innanzi tutto, il rilievo del senatore Li Gotti personalmente non lo condivido, ma, in ogni caso, dichiaro la mia totale totale disponibilità a modificare il testo in modo tale da superare quel dubbio sui cinque anni richiesti come requisito per potersi iscrivere all'elenco dei difensori d'ufficio. In secondo luogo, gli argomenti ora esposti dal senatore Longo mi appaiono abbastanza inconferenti: mi chiedo infatti cosa c'entri il fatto che la Corte costituzionale ha stabilito che i praticanti avvocati non possono assumere la difesa d'ufficio.

all'unanimità si è evidenziato un codice antimafia per cui chi è condannato non può essere inserito nelle liste elettorali,

innanzitutto vorrei che fosse posto ai voti anche l'emendamento 16.204, trattandosi della medesima materia. Presidente, non vorrei aggiungere ulteriori parole a quelle che aveva già così brillantemente speso la senatrice Finocchiaro quando abbiamo illustrato questi emendamenti. Vorrei dire peraltro che è veramente inconcepibile voler confondere la legge con il codice deontologico. Di fronte ad una presa di posizione ingiustificata e grave della maggioranza e anche del Governo, che non vuole far inserire un principio che oggi è passato all'unanimità perfino in Commissione antimafia, resto stupita, non posso che prenderne atto e insisto perché l'emendamento venga approvato.

(testo 2) ha una sua specificità. Il fatto che nel corpo dell'articolo proposto sia previsto comunque di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense» introduce, come già è stato detto in Commissione, un giudizio di attualità: essere di condotta irreprensibile. L'emendamento invece prende in considerazione coloro che abbiano riportato condanne definitive per mafia: sono due cose diverse. L'attualità della condotta irreprensibile non è un mantello largo che copra tutto: si tratta di fattispecie e di previsioni diverse. Noi riteniamo che colui che abbia riportato una condanna definitiva per reati di mafia non abbia titolo per l'iscrizione in un albo dal quale discende anche come conseguenza la possibilità di iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio, ossia l'osservanza ed obbligo della prestazione di un ufficio reso nell'interesse della giustizia. Riteniamo che tra i requisiti richiesti per coloro che possono anche iscriversi nell'albo dei difensori d'ufficio, e quindi nell'elenco dell'albo degli avvocati, debba anche farsi riferimento alle condotte di vita pregresse:

Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è noto come l'elencazione tipica di alcuni reati induca l'interprete a ritenere che il legislatore abbia escluso o ritenuto comunque di minore importanza - e qui si parla dell'iscrizione all'albo degli avvocati - gli autori di altro genere di reato. Da più di un secolo la dizione «condotta irreprensibile» è un mantello estremamente largo, che tra l'altro è stato anche applicato con estrema severità proprio dal Consiglio nazionale forense - di questo penso gli si possa dare atto - ai fini dell'individuazione di condotte anche non ricadenti in una norma penale che comunque non potevano essere considerate irreprensibili. [**Presidenza del vice

Si entra nella logica secondo cui una norma che ha carattere generale e di copertura complessiva diventa esclusivamente una norma manifesto. Ma veramente abbiamo ancora bisogno di queste norme manifesto nel nostro ordinamento? Non si riesce ad avere un ordinamento che reagisca senza bisogno di queste indicazioni di massima,

alla demagogia e al populismo, che non fanno che nuocere complessivamente alla legge.

non fanno ritenere decoroso al Consiglio nazionale forense la permanenza di quell'avvocato nell'albo professionale

farsi strada anche una interpretazione malpensante di questa ostinazione. È una ostinazione incomprensibile.

questo emendamento e i reati che vengono citati, proprio perché riteniamo indispensabile una certa chiarezza, pulizia e trasparenza anche all'interno dell'albo degli avvocati.

previsti anche gli altri gravi reati citati dal Sottosegretario e dal senatore Centaro, quali quelli - ad esempio - di truffa e di appropriazione indebita commessi da avvocati.

la falsa testimonianza, la frode processuale, le false dichiarazioni o attestazioni, la subornazione di testimone, il patrocinio infedele o altre infedeltà del difensore. Ora, se si ritiene che possa essere iscritto e rimanere iscritto nell'albo, e quindi non si debba cancellare, un avvocato macchiatosi con sentenza definitiva passata in giudicato di patrocinio infedele o di altre infedeltà nonché di subornazione, di frode processuale o di tutti gli altri gravissimi reati, non si comprende che cosa si voglia fare di questo ordine.

quello che ora si ripropone, anche con l'intervento del senatore Casson, è una sorta di condanna perenne di colui che ha subito una sentenza di condanna. Siamo di fronte al solito vecchio problema, che si trascina da molti decenni: se la pena abbia un effetto retributivo o di prevenzione speciale. speciale. Se qualcuno è condannato e poi ovviamente, per il tipo di condanna, è escluso dai pubblici uffici perché interdetto a vita, è un discorso. Ma quando un soggetto ha pagato il suo debito - come si dice in forma corrente - o ha avuto addirittura la riabilitazione, siamo in presenza di un cittadino che,

vogliamo ancora continuare a sostenere, com'è stato fatto per molti decenni, che uno che ha subito una sentenza di condanna, come tale debba essere sempre considerato pericoloso per la società? Non credo proprio.

ci può essere una giurisdizione differenziata rispetto alla valutazione della condotta dei singoli iscritti agli albi professionali?

quando non si vuole scrivere qualcosa, la si delega all'autonomia del Consiglio nazionale forense o di chissà chi; mentre quando si vuole scrivere qualcosa lo si fa così puntigliosamente da rendere impossibile

secondo le regole della nostra Costituzione, ha titolo e diritto per tornare ad esercitare l'attività forense. Non possiamo però dire che l'attività forense ha un suo rilievo costituzionale, una sua specificità e che necessita di una specializzazione e di una sua esclusiva e poi

Signor Presidente, raccolgo le indicazioni, sia del senatore Longo sia, soprattutto, del senatore D'Alia. Sarebbe opportuno questo accantonamento. Tra l'altro per questo emendamento già nel precedente passaggio in Aula del Governo ed il relatore mi sembrava avessero dimostrato una qualche disponibilità. Quanto è stato segnalato è sicuramente corretto. Ci sono almeno tre strade: quella di specificare meglio il comma 14, che già prevede la possibilità

considerato che è obiettivo del tutto primario assicurare una regolamentazione volta al corretto contemperamento della tutela dell'avvocato, che si trovi in maternità o in condizioni di allattamento, con un con un andamento spedito dei procedimenti civili, penali e amministrativi cui l'avvocato medesimo prende parte, garantendo altresì il diritto del cliente di farsi assistere dal professionista cui ha conferito il mandato e in favore del quale ha riposto la propria fiducia, impegna il Governo a proporre iniziative legislative volte a consentire che la donna avvocato in stato di maternità possa ottenere a tutela della salute della madre e del nascituro rinvio di udienza qualora nel processo penale sia acquisito il consenso dell'imputato, e della parte offesa, nel processo civile il consenso delle parti e della controparte, e in sede di procedimenti di volontaria giurisdizione, anche del pubblico ministero. In ogni caso, si potranno prevedere appositi istituti per i quali

e il sacramento della confessione praticato dal ministro del culto. Si tratta di un grave problema, che non si può sottovalutare. Ripeto, la soppressione dell'incompatibilità

va esattamente nella direzione opposta di quanto previsto da un emendamento approvato la settimana scorsa, prima che il testo ritornasse in Commissione, che sopprimeva un'incompatibilità.

che era stato approvato quando «invita pertanto il Parlamento a riesaminare con attenzione questo grave e rilevante problema e, in perfetta autonomia dal mondo imprenditoriale» - ma non da quello forense, aggiungo io - «ad eliminare la contestata disposizione».

rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale». Ora, se noi introduciamo

ne deriva un *handicap* negativo, una discriminazione al contrario che noi infliggiamo agli avvocati italiani. È chiaro che, essendo la legge comunitaria una norma

Stiamo introducendo una discriminazione al contrario ai danni degli avvocati italiani. L'avvocato francese, inglese o spagnolo può esercitare la professione anche avendo altrove un rapporto di lavoro *part time*?

*(PD)*. Signor Presidente, lo diciamo spesso, ma questa volta mi auguro veramente che gli avversari, soprattutto i colleghi che sono in grado di seguire e che stanno seguendo con molta attenzione lo svolgersi di questo dibattito, prestino la dovuta attenzione, cominciando dal relatore. Questo emendamento non tende ad escludere nessuno in maniera punitiva, come mi sono sentito dire a proposito di un altro emendamento.

non possa assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3*‑bis*: reati di mafia, terrorismo e reati contro la pubblica amministrazione. Non sfioro minimamente il diritto alla difesa, non c'entra il diritto alla difesa. Egregi colleghi che vi opponete in maniera veramente incomprensibile, abbiamo tre soggetti: la criminalità organizzata (la mafia o le mafie), l'avvocato e il parlamentare. Ho ascoltato con attenzione i discorsi precedenti che riguardavano la possibilità di escludere l'iscrizione. E si parla di una serie di reati PdL)*. Un minimo di attenzione! Parliamo di criminalità organizzata, di mafia: nel nostro Paese questo è un fenomeno tristemente noto e tristemente attuale. Al concetto e al fenomeno della mafia è legato purtroppo nel nostro Paese, e per fatti di grande rilevanza, il connubio, la capacità invasiva e pervasiva del crimine organizzato, che non ha risparmiato nessuno, niente, nessun luogo, nessuna istituzione. Abbiamo avuto persino in questa Aula qualcuno che poi è stato legittimamente e giustamente allontanato e vi era la pervasività, in quella figura, del crimine organizzato. Allora, qui non stiamo parlando di togliere nulla agli avvocati.

mafia. Quello che sto dicendo è tanto vero che siamo in un Paese in cui a distanza di decenni si va a riesumare un cadavere per vedere se è quello del bandito Giuliano. Ma perché tutto questo? Siamo in un Paese dove è accaduto di tutto, dai giorni della Liberazione ad oggi. Allora vi chiediamo di ragionare, di essere sereni. Un processo per mafia in cui si veda l'avvocato parlamentare

Allora, possiamo una volta tanto ritrovarci insieme nella difesa delle istituzioni? Difendiamo l'avvocato! Per motivi anagrafici ho visto un passaggio lungo e faticoso nella figura dell'avvocato, emarginato decenni or sono. Oggi avanza in maniera sempre più prepotente e più dignitosa, assumendo giustamente il ruolo che gli compete. Quindi non vale più dire: ma tanto l'avvocato ha un ruolo diverso da quello del magistrato! Certamente è diverso, ma nondimeno ha pari dignità, e non si può consentire che difenda Provenzano, Riina e compagnia bella nel momento in cui si riveste la carica di parlamentare Perché in questo momento non deve sospendere la sua attività, lanciando un messaggio positivo? Altrimenti, il messaggio sarà negativo: i cittadini saranno indotti a ritenere che il parlamentare,

la figura del parlamentare e quindi la dignità delle istituzioni? Per questo vi invito a ragionare e a votare a favore di questo emendamento. signori del Senato, non mi meraviglio di avere un concetto di avvocato profondamente diverso da quello espresso dal senatore Maritati.

Qui non si riesce a comprendere da parte di qualcuno che all'avvocato penalista - perché credo che l'emendamento sia stato confezionato soprattutto in relazione ai processi penali penali - ci si rivolge quando le cose sono già accadute, tranne casi particolari, come il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione quando ancora il soggetto è in mano ai sequestratori, o per certi fenomeni di reati reati permanenti; ma sono delle nicchie. Che cosa vuol dire? La difesa è assicurata dalla Carta costituzionale come inviolabile; e tanto più è efficace quanto più il soggetto può scegliere chi vuole come suo avvocato. Poi dipende dalla sensibilità di ciascuno accettare o meno, se la causa la conosce, se quella materia la conosce o meno. Però facciamo una proposta, che certamente è provocatoria (d'altra parte se non si fanno le provocazioni in questa sede non vedo dove farle):

Signor Presidente, annuncio il voto contrario mio e della senatrice Poretti, ricordando il lavoro del nostro compagno di partito, già senatore, Piero Milio, che proprio svolgendo la sua funzione di avvocato riuscì a

posso arricchire di una ulteriore considerazione che non si è mai affacciata questo pomeriggio in quest'Aula. La considerazione è su quel diritto alla difesa

nella scelta del proprio difensore che è sovraordinato ad ogni esigenza, pur condivisibile ovviamente, di sospetto sulla professionalità dell'avvocato. *(Applausi dal Gruppo*

messo da parte, in maniera, io ritengo, erronea e superficiale, nel senso di una mancanza di sereno approfondimento. Mi chiedo: che cosa ha a che fare la libertà dell'avvocato, la sua indipendenza, la scelta libera di un difensore, che lo stesso decida di scendere in politica, venga eletto legittimamente e nominato presidente di una Regione?

qualcosa possa accadere o qualcuno possa pensare che le cose non vadano regolarmente in un processo e che gli altri avvocati osservino tale sbilanciamento? Continuo veramente a rimanere attonito davanti all'inerzia di molti di voi, che certamente non possono abbracciare questa filosofia del tanto peggio, tanto meglio per qualcuno. Qui stiamo lavorando per garantire gli interessi non di una categoria ma di un numero ristrettissimo di personalità o persone che diventano potenti con il potere che esercitano. È mai pensabile che questo possa accadere anche con gli assessori regionali, cioè con gente che oggi ha un enorme potere di gestione e di conferimento di incarichi? tutto ciò deve passare perché altrimenti si incide sulla libertà dell'avvocato? Ma nel periodo in cui liberamente abbiano scelto di diventare rappresentanti delle istituzioni, che lo facciano a tempo pieno. In questo Paese non possiamo andare avanti.

dovrebbe essere patrimonio di tutti noi. Non è eticamente accettabile che chi ricopre determinate cariche dello Stato o della Regione eserciti un'attività liberale importantissima e degna di massimo rispetto, qual è quella dell'avvocato. Stiamo approvando una legge nuova; fermatevi,

il parere è favorevole a condizione che venga riformulato nel senso: che venga espunta la lettera

sull'operazione che viene compiuta rispetto ad una professione che si definisce liberale. L'esercizio di una professione liberale viene assoggettata a determinati requisiti vincolanti, per cui un'attività non continuativa dà luogo alla cancellazione dall'albo di una persona che ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e che successivamente si iscrive. Al di là della

di questo disegno di legge, in cui è stato eliminato il riferimento all'attività abituale e prevalente - chiedo seriamente se sia possibile che il Consiglio nazionale forense decida la cancellazione di un libero professionista senza incorrere in violazione di norme costituzionali inderogabili. Il senso dell'emendamento è questo, è un richiamo a questi profili. Per questo si vogliono rimettere

dopo una procedura attenta, valuterà «se possano essere configurate, nell'interesse pubblico» ma anche nell'interesse «della libera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all'albo, indipendenti da violazioni disciplinari conformi a principi di pari opportunità e non discriminazione,» (ricordo che il diritto discriminatorio ormai fa parte del nostro ordinamento) «nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta costituzionale, tenendo altresì conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità

prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo». Dunque, dal momento che il contraddittorio è previsto, vorrei che venisse meglio specificato

la domanda è sicuramente tendenziosa. Mi dispiace, ognuno legge le norme e ne trae le conseguenze.

vertendo in materia di diritti costituzionalmente protetti, qual è il contraddittorio, era di rilievo il suo argomentare in ordine a questo articolo. Avendo quindi colto parzialmente le ragioni di argomentazioni serie, mi ero permesso, in forma probabilmente irrituale, di sollecitare un'interlocuzione: so che il Regolamento non lo consente, però in altre occasioni ciò comunque

Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza» - cioè, gli ordini degli avvocati, composti dagli avvocati, hanno come loro finalità prevalente la tutela dell'utenza «e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto» - ovviamente - «delle e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia». Il cuore di tutta la legge alla fine è qui. Gli ordini e il Consiglio nazionale forense cosa sono? Sono associazioni associazioni che in qualche modo tutelano gli iscritti e gli associati, oppure no, come recita il testo della legge? Sono enti pubblici, che addirittura dovrebbero in primo luogo tutelare chi si rivolge agli avvocati? Credo che questo aspetto davvero debba essere chiarito e, per quanto ci riguarda, presentiamo un emendamento

ordini sono associazioni di categoria a carattere privatistico che tutelano gli interessi degli iscritti. Ciò va davvero incontro a quello che dovrebbe essere la libera professione, costituita da liberi professionisti

Probabilmente si potrebbe trovare una soluzione; infatti, nel momento in cui si dichiara che si finanziano tutti con contributi privati e hanno autonomia finanziaria, perché mai perché mai dovrebbero essere enti pubblici, ancorché non economici, e quindi sottoposti alla vigilanza dello Stato? Il punto è proprio questo.

visto che ci si finanzia con contributi interamente privati, viene fatto salvo sia il principio della finalità, assolutamente importante, sia la questione relativa alla copertura delle eventuali spese, perché, ancorché

L'Ordine forense persegue più finalità, come è proprio di molti ordini professionali: sia la tutela di carattere interno riguardo all'osservanza delle norme deontologiche ed anche l'esercizio del potere disciplinare, sia i rapporti con i terzi, con l'esterno, sia, soprattutto, quella funzione di garanzia verso l'utenza, di tutela della credibilità nei confronti dei clienti, che abbiamo sottolineato in più passaggi. Proprio per questo scopo è stato concepito l'emendamento 23.204 della Commissione, che sintetizza tali esigenze.

di un pluralismo sociale che è il cuore delle democrazie moderne: cioè proprio l'associazionismo che viene investito di responsabilità e che le assume nei confronti dei terzi. È una funzione pubblicistica che, non a caso

Questa vigilanza è giustificata dal rilievo pubblicistico delle sue funzioni. Queste sono le ragioni per le quali è giusto che il testo resti quello che è, con la modifica di cui all'emendamento 23.204, che viene incontro alle queste esigenze o perplessità che avete giustamente manifestato.

Credo che la notte potrebbe portare consiglio e, pertanto, se potessimo rinviare a domani mattina il tutto, sarebbe la cosa migliore. PRESIDENTE. Il relatore vuole accantonare l'emendamento

abbiamo lavorato alacremente, per cui potrei anche non oppormi. La ragione per la quale l'Ordine resta

Ha una sua funzione pubblica di tutta evidenza: è l'unico sopravvissuto ai cambiamenti e alla Costituzione. Questa è una ragione fondamental: non possiamo rendere privata l'amministrazione della giustizia, sia pure giustizia domestica.

rivolta al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e finanze. Non infierisco sull'inerzia del Governo a questo proposito, però sottolineo che è trascorso più di un anno e ancora non c'è stata risposta su un argomento e un problema non di scarso profilo: le modalità di utilizzo dei buoni pasto, che sono buoni di valore predefinito concessi dai datori di lavoro ai dipendenti in sostituzione della mensa aziendale. Nella mia interrogazione chiedevo di sapere se il Governo intende intervenire per adeguare al costo della vita il valore dei buoni pasto, perché è molto tempo che non vengono adeguati, e per vengono adeguati, e per impedire che le gare al massimo ribasso si svolgano in modo tale da penalizzare esercenti e consumatori finali considerato che le commissioni per gli esercizi che ritirano i buoni pasto arrivano cento, e di conseguenza, il valore facciale del buono subisce un taglio secco. Il problema, dicevo, non è di scarso profilo: è di assoluta attualità, in un momento di crisi come l'attuale.

non offre alcuna possibilità di controllo e di sanzione nei confronti di coloro che non rispettano la norma. Auspico, quindi, che entro breve sia data risposta a questa interrogazione.

a recepire il decreto ministeriale che appunto si occupa di questo provvedimento. Cosa comporta il mancato recepimento di questa disposizione? I reclusi della Regione Sicilia non godono degli stessi servizi, dello stesso livello di assistenza degli altri reclusi in Italia. Non solo: questo mancato recepimento determina

Come lei sa, signor Presidente, nella nostra Regione siciliana, si sono verificati fatti di malasanità penitenziari molto gravi; anche nella sua Messina, così come nella mia Catania. Tutti questi fatti sono stati regolarmente segnalati e portati all'attenzione dell'opinione pubblica, ma segnano, purtroppo, ove ve ne fosse ulteriormente bisogno, una crisi di un settore, che ovviamente è aggravata dal fatto che la Regione non ha ancora provveduto a compiere il proprio dovere. Le motivazioni che la Regione formula a questo proposito riguardano la Commissione paritetica Stato-Regione relativamente ai costi che questo trasferimento di competenza determinerebbe. Io ritengo che questa osservazione sia del tutto pretestuosa perché il decreto è del 2008 (sono passati oltre due anni)

che il mancato recepimento di questo decreto possa determinare un discrimine così grave, in violazione del diritto alla salute, contenuto nella Costituzione italiana, tanto da non

Signor Presidente, vorrei rilevare che oggi è avvenuto un fatto importante: Susanna Camusso è stata eletta segretario generale della CGIL, il più grande sindacato italiano. Questo fatto è estremamente importante, perché Susanna Camusso assume questo incarico in un momento delicato per la situazione economica

Non è la prima volta che una donna è chiamata a condurre un sindacato importante: ricordo che nel 2002 Renata Polverini è stata eletta segretario generale dell'UGL. PRESIDENTE. Allora diventerà anche lei presidente di qualche Regione.

auguriamo. Così come oggi sono arrivate le congratulazioni del presidente della Camera Gianfranco Fini al nuovo segretario generale, voglio esprimere a e le congratulazioni da parte di tutto il Gruppo di Futuro e Libertà per l'Italia.

oltre ai problemi che ordinariamente si trovano nelle istituzioni carcerarie del nostro Paese, come il sovraffollamento e le problematiche di carenza di organico, è in atto una situazione specifica che credo richieda una risposta in tempi rapidi. c'è una scuola per geometri che viene frequentata anche da detenuti di altri istituti di pena. Questa scuola, da tempo, insieme ad un'altra attività che poi dirò, consente di diplomare delle persone, consente quindi loro una possibilità di alternativa una volta uscite dal carcere, e ha sempre funzionato.

poiché con il provveditorato non ci sono più state ore a disposizione, non sono state più confermate né la scuola per odontotecnici né quella per geometri. È evidente che, con le problematiche presenti nelle strutture carcerarie e il sovraffollamento, la possibilità di avere un'istruzione intanto è, senza scomodare la Costituzione, sicuramente coerente con le disposizioni costituzionali che prevedono per chi è in espiazione